In quello stesso giorno sono state convocate le Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio per iniziare l'esame del provvedimento nel merito. il relatore per la 1a Commissione, senatore Pastore, che ringrazio, ha riferito sul decreto, soffermandosi diffusamente sul suo contenuto, nonché sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, mentre il relatore per la 5a Commissione, senatore Massimo Garavaglia, che ringrazio, rimettendosi alle considerazioni svolte dall'altro relatore, si riservava di intervenire in replica al termine della discussione generale. Nel pomeriggio di quello stesso giorno, 17 marzo, si è svolta la discussione generale. Nella lunga seduta delle Commissioni riunite sono intervenuti i senatori Vitali, Il dibattito è stato dunque molto articolato ed intenso. Gli aspetti sui quali si sono concentrati gli interventi Gli aspetti sui quali si sono concentrati gli interventi del senatore Vitali e poi dei senatori dell'opposizione hanno riguardato, in primo luogo, la lamentata assenza di organicità degli interventi contenuti nel decreto. In particolare, essi hanno evidenziato una contraddizione tra la legge di delega in materia di federalismo fiscale e le norme contenute in molteplici recenti misure adottate dal Governo, che sarebbero ispirate ad una logica di tipo centralista, ritenuta in contrasto con i princìpi autonomisti. Altri rilievi critici, formulati non solo da senatori dell'opposizione, hanno riguardato la riduzione del numero degli amministratori locali: è stato sottolineato che, a fronte di un risparmio modesto, verrebbe ridotta la rappresentanza e la capacità di governo locale, fattore essenziale per la vita della democrazia e per il funzionamento dei servizi per i cittadini. Rilievi critici sono stati espressi anche sulla norma che esclude dal saldo finanziario, rilevante ai fini del Patto di stabilità, le spese sostenute dagli enti locali per i cosiddetti grandi eventi: in proposito, è stato paventato il rischio di un indiscriminato Il senatore Morando, in particolare, ha concentrato il suo intervento sulle ricadute negative di carattere finanziario, osservando che le disposizioni contenute nel decreto farebbero venire meno le condizioni del risparmio atteso, con effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. senatore Malan ha manifestato il suo apprezzamento per le norme che determinano una efficace razionalizzazione della finanza locale, mentre il senatore Benedetti Valentini ha osservato che il carattere limitato degli interventi previsti nel decreto-legge dipende proprio dallo strumento legislativo prescelto, essendo la decretazione d'urgenza un mezzo inadeguato per interventi di carattere strutturale più approfonditi. Nel riconoscere il merito dell'Esecutivo di aver iniziato un audace percorso di cambiamento, il senatore Benedetti Valentini ha espresso, tra l'altro, il suo apprezzamento per le norme volte a ridurre il numero dei consiglieri e degli assessori. Sostanzialmente condivise sono state invece le misure a favore dei territori colpiti dal sisma in Abruzzo. Giovedì 18 marzo le Commissioni si sono di nuovo riunite per le repliche dei relatori e dei rappresentanti del Governo, nonché per l'esame dei circa 200 emendamenti presentati. Il relatore Pastore ha ricordato che non sarebbe stato possibile introdurre in un decreto-legge norme di carattere ordinamentale di natura organica. Il provvedimento d'urgenza ha invece inevitabilmente una portata limitata, volta a rendere più equilibrati gli interventi di contenimento dei costi della politica approntati con la legge finanziaria per il 2010. Il relatore Massimo Garavaglia, dopo aver espresso la sua condivisione circa l'opportunità che per il futuro la qualifica di grande evento sia riservata solo a poche iniziative di particolare rilievo, ha sottolineato la necessità di limitare la proliferazione di enti consortili che hanno dimostrato, nella maggioranza dei casi di non essere efficienti e di dar luogo ad un inopportuno aggravio dei costi per il funzionamento degli enti locali. Il vice ministro Vegas, nell'apprezzare il contenuto di alcuni interventi, in particolare in riferimento al Patto di stabilità, ha rilevato che, in sede di attuazione del federalismo fiscale, sarà possibile procedere con le opportune modifiche, ma ha pure, nello stesso tempo, rilevato la necessità di una rigorosa applicazione del Patto stesso per non oltrepassare i limiti del fabbisogno e per evitare così sanzioni da parte dell'Unione europea. Il ministro Calderoli, nel replicare puntualmente ai numerosi interventi in discussione generale, ha ribadito gli auspici del Governo perché le riforme organiche di natura ordinamentale possano procedere quanto più possibile celermente. Ha ricordato, in proposito, che il cosiddetto codice delle autonomie, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri dopo lunga attesa, senza il parere della Conferenza Stato-Regioni, benché sia stato presentato alla Camera nel mese di gennaio, è ancora ad uno stato iniziale dell'esame in Commissione nell'altro ramo del Parlamento. Dopo le repliche, nel passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, sui quali il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario, per due volte consecutive è stata constatata la mancanza del numero legale al momento della votazione sul primo emendamento.

giorno e per i giorni successivi, nonché considerando la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea per la giornata di oggi, ho dovuto rilevare che non vi erano le condizioni per concludere la trattazione del disegno di legge in sede referente in tempo utile per la discussione in Aula. Le Commissioni riunite hanno concordato in tal senso. Desidero però sottolineare che le Commissioni riunite in sede referente - come si evince da ciò che ho poc'anzi riferito - hanno comunque svolto un'ampia ed approfondita discussione su ogni aspetto del decreto e sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe senatrici e colleghi senatori, com'è noto l'articolo 77 della nostra Costituzione prevede che i decreti-legge emanati dal Governo debbano avere i presupposti di necessità e di urgenza. La legge n. 400 del 1988 stabilisce poi che gli atti assunti in forza di questo articolo della Costituzione debbano contenere nel preambolo l'indicazione delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione. Nel preambolo del decreto-legge oggi al nostro esame viene

In questo decreto vi sono alcune norme che corrispondono a queste esigenze - in modo particolare quelle riferite alla proroga al 2011 della riduzione del numero dei componenti degli organi elettivi comunali e provinciali - ma ve ne sono altre che non hanno assolutamente questo carattere. Ancora una volta, quindi, si utilizza il veicolo dei decreti-legge per sopperire alla mancanza di volontà da parte dell'Esecutivo di favorire la funzione legislativa autonoma del Parlamento. Siamo ancora di fronte a quell'espropriazione del ruolo del Parlamento che più volte abbiamo denunciato. Pertanto, con la scusa dell'impossibilità di portare avanti disegni di legge ordinari, si riempiono i decreti-legge di norme che non hanno minimamente il carattere di necessità e di urgenza.

Su questo ci potrebbe anche essere la possibilità di sviluppare una discussione, che potrebbe portare anche ad esiti condivisi, ma dovrebbe essere fatta propriamente, e cioè senza usare lo strumento del decreto-legge. È evidente che per questo non c'è alcuna urgenza. Questo vale anche per l'articolo 1, comma là ove si stabilisce una modalità attraverso la quale le funzioni del difensore civico comunale vengono attribuite a quello provinciale, e si escludono i bacini imbriferi montani dalle soppressioni di organi intermedi previste dalla legge finanziaria del 2010. La stessa cosa vale poi per l'articolo 1, comma 1-*quinquies*, là ove si stabilisce la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale ad un anno di scadenza dall'entrata in vigore di questo decreto. potete vedere, si tratta di materie di carattere ordinamentale, sulle quali assurdamente il Governo è intervenuto con un emendamento alla legge finanziaria del 2010,

di rivedere alcune di queste norme, ad un mese di distanza dall'approvazione della finanziaria il Governo ha presentato un decreto, per di più infilandoci dentro norme che nulla hanno a che vedere con i requisiti di necessità e di urgenza. Si è quindi, volutamente, impedito al Parlamento di discutere di quella carta delle autonomie locali che noi, Gruppo del Partito Democratico e Gruppi di opposizione, da 10 mesi che venga portata all'attenzione delle Camere, cioè da quando votammo, in modo definitivo in quest'Aula, la legge sul federalismo fiscale. Il ministro Calderoli ci ha detto che solo recentemente è stato possibile pervenire a una proposta definitiva presentata dal Governo alle Camere. Bene, allora che si discuta su quel testo, che si eviti d'intervenire in questo modo, con leggi finanziarie o decreti-legge che non rispondono minimamente ai criteri previsti dalla Costituzione e che si affronti nel merito quel tema. Noi abbiamo molte cose da dire. Siamo sicuramente d'accordo per una riorganizzazione di tutto il sistema degli enti locali, compresa anche la riduzione del numero dei componenti di vari organismi, ma siamo soprattutto d'accordo per una riduzione delle funzioni dei Ministeri centrali, misura sulla quale la proposta del Governo non dice una parola. Vorrei invitare i colleghi della Lega a prestare qualche attenzione in più su questi temi, perché da un po' di tempo mi sembrano molto distratti.

perché bisogna tener conto delle competenze legislative delle Regioni, anche se su questo tema (e non da ora) noi siamo favorevoli ad una forte semplificazione di tutti questi organismi di secondo grado.

i commi dal 4-*quinquies* al 4-*novies* dell'articolo 4, che prevedono deroghe al Patto di stabilità interno. Ora, sia chiaro noi, come Gruppo del Partito Democratico, abbiamo di nuovo presentato qui tutta la serie di emendamenti relativi al Patto di stabilità interno, già presentati in sede di discussione della legge finanziaria. Noi crediamo, infatti, che quella sarebbe stata una ragione per intervenire con decreto, per consentire effettivamente ai Comuni di avere maggiore elasticità di spesa di spendere risorse a loro disposizione in un momento di fortissima crisi economica e sociale come questa. Su questo tema, però, Governo e maggioranza non hanno detto una parola. Hanno, invece, introdotto una serie di deroghe molto limitate, una delle quali grida vendetta: luogo, perché non è assolutamente possibile prevedere quanto tale deroga costerà alle casse dello Stato (e, quindi, essa è sicuramente in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione);

anche alla luce delle indagini giudiziarie che coinvolgono il sottosegretario Bertolaso e vedono il suo braccio destro, Angelo Balducci, agli arresti domiciliari, sarebbe stato necessario, da parte del Governo, quantomeno attenersi a un criterio di sobrietà Invece, ancora una volta, viene qui introdotto il concetto di grande evento, come strumento per derogare dal Patto di stabilità interno. È chiaro che vi sono eventi per i quali è giusto derogare,

Qui s'introduce di nuovo la necessità per i Comuni, se vogliono derogare dal Patto di stabilità interno, di presentarsi dal Governo e di chiedere in ginocchio di denominare grande evento una qualunque manifestazione che si svolga nel loro territorio. Vorrei però qui ricordare che, attraverso questo decreto del 2001, da allora ad oggi sono stati dichiarati grandi eventi ben 45 manifestazioni. Bene, alcune di queste avevano davvero quel carattere ma non dovevano essere poste sotto la responsabilità della Protezione civile. Noi chiediamo, infatti, che questa limiti la propria competenza esclusivamente alla calamità naturale e, per il resto, che alla pubblica amministrazione quegli strumenti di efficacia ed efficienza che è possibile darle e che consentano di evitare la vergogna della deroga costante dagli strumenti legislativi. Tra i grandi eventi ricordo anche

che con questo criterio qualunque comune può proporre al Governo di trasformare in un grande evento una manifestazione ordinaria in questo modo, e solo in questo modo, grazie

di respingere questo decreto-legge. Ma vi sono tanti altri motivi per chiedere al Senato di non procedere alla discussione perché palesemente in violazione dell'articolo 77 della Costituzione che richiede veri presupposti di necessità ed urgenza per poter procedere.

di affrontare questa campagna elettorale in un quadro normativo certo, di aprire dunque le nuove consiliature in un quadro normativo definito e di provvedere anche, come è tradizione della nostra esperienza parlamentare, ad affrontare le tematiche di bilancio con interventi finanziari che riguardino gli enti locali che devono provvedere in merito. Mi sembra che le osservazioni del collega Vitali non riguardino tanto l'impianto originario quanto le modifiche apportate dalla Camera, che non sono

che non confligge con i presupposti formali necessari per l'emanazione del decreto-legge. Si tratta di intervenire su figure

per rendere più efficaci, efficienti e complessivamente valide le disposizioni che la finanziaria in quella fase ha introdotto. Ricordiamoci anche che le elezioni degli enti locali sono state anticipate rispetto al termine ordinario,

alla sussistenza dei presupposti d'urgenza in quanto la soppressione degli ATO decorrerebbe tra un anno, faccio presente che l'anno di tempo è stato concesso proprio perché in materia intervengano gli organi regionali con proprie disposizioni, in modo da rappresentare il modello di gestione di quei servizi nella maniera che le Regioni riterranno più appropriata. Tra l'altro, consentitemi un'ultima riflessione. Questo Questo decreto-legge, con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, è di accompagnamento verso l'attuazione del federalismo fiscale e segna, insieme alle disposizioni contenute in finanziaria, un elemento ben preciso,

ai costi e alle scelte del territorio stesso. Lo Stato si libera dal dover assistere questi organismi e attribuisce alle Regioni e alle autonomie locali una piena responsabilità,

e necessità e che rispecchino l'obiettivo politico che il centrodestra condivide e che ci auguriamo anche il centrosinistra possa condividere non solo a parole ma anche nei fatti.

Presidente, onorevoli colleghi, questo decreto-legge, che ha l'obiettivo finale di rivedere i livelli di governo

che punti sulla specializzazione degli enti locali, il Governo ha pensato di procedere ancora una volta secondo la consueta logica dei compartimenti stagni, introduce una serie di criteri che creano differenze e disomogeneità

di criteri che creano differenze e disomogeneità tra i livelli delle autonomie locali che, se questo decreto dovesse diventare legge, non sarebbero più nella condizione di svolgere funzioni amministrative orientate secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti dall'articolo 118 della Costituzione, che - è il caso di ricordarlo a tutti - recita: «Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane,

attraverso il ruolo dei vari riferimenti crea una condizione di responsabilità dei vari livelli istituzionali. si recupera per favorire «l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà» Si ignora, dunque, o si finge di ignorare, che Comuni, Province, Regioni, Città metropolitane e Stato sono sullo stesso livello di rappresentanza democratica. Se questa è la premessa, ne consegue che è inutile, a meno che non si voglia confondere ulteriormente il quadro, tentare di proiettare le disposizioni di questo provvedimento nel quadro del federalismo fiscale

Altro che federalismo, ministro Calderoli! Questo decreto si configura, piuttosto, come un pasticcio, che penalizza le autonomie locali, a partire dai Comuni piccoli, che vengono considerati solo come una zavorra economica, una fonte di spreco, senza rendersi conto del ruolo di rappresentanza di primo livello dello Stato. E il Governo come pensa di intervenire? Tagliando in maniera indiscriminata il numero dei consiglieri e degli assessori, senza tener conto del fatto che tali riduzioni possono pregiudicare l'efficacia e la capacità la capacità di rappresentanza dell'amministrazione locale. Resto convinto che un più largo numero di politici, di chi ha passione civile, nella grave crisi che attraversa la nostra società, può dare un contributo determinante al miglioramento della gestione delle amministrazioni locali, anche attraverso una maggiore specializzazione del lavoro assessori e un più articolato ventaglio di competenza dei consiglieri, quindi delle assemblee. A mio avviso, sbandierare la volontà di ridurre il numero di consiglieri e assessori è proprio di chi vuole fare facile demagogia, sfuggendo alla responsabilità e al necessario impegno per affrontare la questione seriamente e in maniera complessiva. E continuiamo con questa assurda demagogia di svuotamento delle assemblee e delle rappresentanze democratiche. Il Governo interviene in modo scomposto in una materia che richiede attenzione, rispetto per le istituzioni e le comunità e altissimo senso dello Stato. E mi pare di capire che la maggioranza non sia neanche compatta nel sostenere il disegno di legge, parziale e carente di una visione complessiva della questione e del senso di governo dei vari livelli di rappresentanza dello Stato. Non è servito forse a coprire le divisioni il ricorso al voto di fiducia alla Camera? Per la trentesima volta in due anni, un decreto-legge passa con la fiducia: è la prova dell'incapacità della maggioranza di assumere provvedimenti di interesse generale. Altro che federalismo fiscale!

sconfessando, in tal modo, l'operato dell'Esecutivo (oramai momento ricorrente in tutte le espressioni dei vari decreti-legge di questo Governo). Del testo originario è rimasto ben poco: quello su cui ci è chiesto il voto è un maxiemendamento interamente sostitutivo del provvedimento stilato dal Governo in poco meno di un mese. Salvo poi accorgersi degli svarioni e intervenendo non una, non due neanche tre, ma quattro volte per cambiare posizione, senza un disegno complessivo. Le proposte introdotte nella finanziaria 2010 sugli enti locali si discostano da quanto l'Esecutivo ha previsto nella Carta delle autonomie. Si è mai visto che un Governo smentisca se stesso? Berlusconi è capace di tutto, anche di questo. Ebbene, su questo decreto-legge è accaduto: esso si basa, infatti, sulla proroga della quasi totalità delle proposte inserite nella finanziaria, spostata al 1° gennaio 2011. Tutto ciò dimostra, se ve ne fosse ancora bisogno, che non si può condividere la conversione in legge del presente decreto, che non fornisce le risposte attese e pure necessarie sul piano del riordino dei livelli di governo e della redistribuzione delle competenze amministrative sul territorio. I Comuni, soprattutto quelli piccoli, rappresentano il nerbo del tessuto istituzionale e democratico del nostro territorio e la prima interfaccia tra lo Stato e i cittadini. Non è pensabile che essi vengano continuamente smantellati, svuotati. Ne va della tenuta democratica del nostro Paese, specialmente nelle aree a rischio di alta criminalità organizzata, come quelle del Mezzogiorno. Fino a quando si penserà di intervenire su questioni come queste con una visione verticistica, intrisa di populismo ma priva del rispetto che si deve alle istituzioni ed allo Stato, non si affermerà un cambiamento reale del Paese. Serve una riforma complessiva e articolata, che punti a migliorare l'efficienza e l'efficacia degli enti locali, con l'obiettivo di intercettare l'interesse di tutti e non di fare, ancora una volta, propaganda agli interessi di pochi o di chi oggi rappresenta, più che lo Stato e gli interessi generali della comunità, l'interesse privato della propria azienda senza avere senso dello Stato, né a cuore la difesa della democrazia.

Camera. Con questo provvedimento siamo giunti ad un rimedio peggiore del male, e c'è da dire che l'intero percorso sugli enti locali da parte del Governo ci è parso altalenante, incerto, confuso e in qualche caso perfino contraddittorio.

quando ci apprestammo all'esame dei provvedimenti sul federalismo, ritenendo che la definizione delle funzioni e delle competenze fosse prioritaria ad affrontare quello stesso argomento; ma purtroppo in quella sede si fu pressati dal tema del federalismo, prima ancora della definizione delle competenze e di una riforma organica degli enti locali. ha provveduto ad intervenire sugli enti locali in modo molto contraddittorio: prima con la Carta delle autonomie (ripeto, da noi sollecitata), poi con la finanziaria 2010, che contraddiceva alcune questioni poste nella Carta delle autonomie, ed infine con il decreto, che correggeva alcuni errori, abbastanza grossolani, presenti nella stessa finanziaria.

si è cambiata idea su molti degli aspetti presenti nei provvedimenti che ho qui citato. Sembra quindi di riscontare una visione sicuramente non omogenea sugli enti locali, una scelta sbagliata che lede almeno tre principi: il principio della leale collaborazione tra Stato ed enti locali, quello dell'autonomia statutaria, sulla quale si interviene pesantemente, e, ancora, il principio dell'autonomia organizzativa. Dal punto di vista della leale collaborazione, cosa dire sul fatto che, mentre gli enti locali discutevano al tavolo con lo Stato sul tema della riforma e della Carta delle autonomie, il Governo stralciava alcune misure per introdurle nella finanziaria? E ancora, sull'autonomia statutaria, si è leso tale principio andando ad incidere fortemente sull'organizzazione statutaria degli enti relativamente alle circoscrizioni si elimina la figura del direttore generale, contravvenendo a tutte le questioni roboanti spesso poste sulla riforma della pubblica amministrazione, sugli obiettivi di efficientizzazione della stessa e della cosiddetta managerialità. Potremmo dire che questo Governo contraddice l'operato dei suoi Ministri, e che un Ministro smentisce l'altro, mentre intanto ci si orienta tutti a tagli ragionieristici che fanno solo propaganda sul costo della politica che incontrano forse qualche favore elettorale, a cominciare dai più piccoli, dai meno costosi, senza guardare ai moltissimi ed onerosi costi costi che si generano per molte cariche pubbliche e per apparati centrali, non solo politici e di rappresentanza. Cosa dire poi di tutto il percorso di tanti enti che andrebbero disboscati e che il Governo Prodi aveva iniziato ad esaminare con una certa capacità di analisi su quanto questi fossero del tutto inutili e molto spesso costosi per la collettività? Non vi è una vera credibilità, un vero programma di revisione, di riforme, di riconversione della spesa, di riduzione dei costi, certo, ma anche di qualità della spesa. Intanto gli enti locali sono in ginocchio, a partire dalla sciagurata decisione sull'ICI, al tema dei trasferimenti, al dilapidare dei fondi FAS a cui abbiamo assistito. I cittadini e le imprese sono in difficoltà. Abbiamo fatto numerose proposte per far sì che venissero pagate le opere già previste e coperte da investimenti, quelle finanziate nonché quelle cofinanziate anche dai fondi europei.

questi costi dovranno necessariamente trovare compensazione attraverso o una rimodulazione delle restanti voci o un incremento delle entrate degli enti in questione. Ancora una volta, quindi, si scarica tutto sugli enti locali, sui cittadini e sui servizi. Ma quale fiducia avete posto alla Camera ed avete chiesto ai cittadini? La verità è che voi avete una sfiducia molto profonda verso alcuni principi fondamentali ed assetti istituzionali del nostro Paese, che vi porta ad alcuni provvedimenti davvero improvvisati.

per riformare occorre cooperare, ascoltare, collaborare, decidere in modo autorevole, creare un percorso di merito non improvvisato né autoritario. La fatica del Governo non è solo comando: è ardua e difficile, deve fare i conti con la complessità del Paese, certamente con le sue arretratezze e lentezze, perfino con la pesantezza della politica, ma la sfida si vince solo con l'autorevolezza con l'autorevolezza di chi riesce a far andare avanti il Paese, fa i conti con tutto ciò ed ha il coraggio di fare le riforme. Per il momento l'Italia è ferma e resta molto indietro, scarica ancora una volta sugli enti locali e sui cittadini l'incapacità di affrontare qualitativamente alcune riforme di fondo di cui il Paese avrebbe bisogno.

Presidente, onorevoli colleghi,

perché siamo schiacciati dalla consapevolezza che i tempi di conversione in legge non consentono la modifica del disegno di legge di conversione: ci sembra quindi più utile provare a suggerire al Governo un atteggiamento costruttivo per rimediare ai danni obiettivi che il provvedimento in esame ha in sé. I temi fondamentali sono quelli che riguardano i servizi pubblici, in particolare rifiuti e acqua, e la commistione, terribile, tra le calamità naturali e i grandi eventi. Sul primo punto, il comma 1-*quinquies* dell'articolo 1 stabilisce la soppressione entro l'anno delle Autorità d'ambito territoriale,

innovazione, che è incoerente, deve essere valutata nelle sue conseguenze dirette: il Governo deve essere impegnato a studiare e a tenere sotto controllo, in coordinamento con gli enti territoriali competenti, gli effetti applicativi e le ricadute su elementi fondamentali come la risorsa idrica e la gestione dei rifiuti urbani, soprattutto in riferimento alle tariffe che ricadono sui cittadini. Ora, il provvedimento prevede una fase transitoria fino al subentro di nuovi soggetti individuati con legge regionale, ma sovrappone questa nuova scelta alla fase attuativa della riforma - assai controversa - sui servizi pubblici, introdotta con la legge n. 133 del 2008 e la legge n. 166 del 2009, che ha prospettato una sorta (speriamo sia solo una sorta) di privatizzazione dell'acqua. Non è chiaro quali effetti possano esservi sulle gare da parte di norme che prevedono il passaggio a soggetti individuati con legge regionale: bisogna considerare, infatti, che indire una molteplicità di gare in ambito e per ambito potrebbe virtualmente garantire l'esercizio della concorrenza. Al contrario, una ventina di gare potrebbero finire per sottoporre i Comuni a tentazioni monopolistiche o oligopolistiche. Qui il pessimismo è d'obbligo; ma di questo aspetto la legge non si occupa, lasciando invece nel vuoto normativo l'intera questione. Sarebbe invece necessario che il Governo, sempre d'intesa con le istituzioni competenti, assicurasse il coordinamento della disposizione con la normativa vigente al fine di garantire che sia nella fase transitoria sia nella fase attuativa il servizio di gestione integrata dei rifiuti dell'acqua risponda agli obiettivi fondamentali di tutela ambientale e agli standard qualitativi ottimali del servizio, secondo il principio di accessibilità universale. Questo per quello che riguarda la questione della commistione indebita tra calamità naturali e grandi eventi, bisogna rilevare che, dopo le polemiche dell'ultimo periodo e i solenni impegni presi dal Governo in relazione al Patto di stabilità, il decreto in esame equipara le spese per i grandi eventi a quelle per calamità naturali. Ebbene, l'operazione è sì limitata ai trasferimenti statali e alle spese da questi finanziate, ma per le spese sostenute dai Comuni con risorse proprie queste restano rilevanti, per questo aspetto, anche se sono collegate ai grandi eventi. In pratica, abbiamo Comuni penalizzati e confusione tra grandi eventi ed emergenza. Grandi eventi, non dimentichiamolo, che spesso si configurano come colossali operazioni di spettacolo propagandistico: qualche volta abbiamo dovuto assistere - nel caso dell'Aquila abbiamo soffrendo assistito - al fatto che un'emergenza di carattere naturale è stata anche trasformata in una colossale operazione di spettacolo propagandistico. Il taglio dell'ICI ha notoriamente impoverito i Comuni, i quali devono anche gestire le conseguenze della sentenza n. 238 del 2009 della Corte costituzionale che, in modo tecnicamente ineccepibile,

cosiddetto federalista, invece, lascia indifesi i Comuni proprio di fronte a vuoti di bilancio causati sia dalle sue scelte, sia, di fatto, da questa sentenza (che però, sotto il profilo tecnico, è ineccepibile). Va ricordato che anche la dottrina costituzionale ha denunciato l'espansione crescente delle ordinanze di protezione civile, allargate ai campi più inverosimili. La norma in esame, relativa alla questione dei grandi eventi e delle calamità naturali, può avere senso solo per le vere calamità naturali, ma non certo per i grandi eventi.

rivolgiamo anche un ulteriore invito al Governo affinché provi, se ci riesce, a ricondurre nel corretto alveo ordinamentale l'impiego delle ordinanze di protezione civile per quanto riguarda i cosiddetti grandi eventi, al fine di assicurare la massima trasparenza dei finanziamenti pubblici - come dicevo - secondo un impegno che apparentemente è stato già assunto, ma che in realtà non è ancora stato mantenuto dal sottosegretario Bertolaso.

a Palazzo Madama. A lui rivolgiamo il nostro benvenuto e il nostro saluto, nello spirito di amicizia e collaborazione tra i nostri due Paesi reso più forte dalla comune appartenenza all'Unione europea.

n. 2071 rappresenta un ulteriore esempio dell'incapacità del Governo di legiferare in modo organico per un reale processo di riforma del sistema istituzionale. Ancora una volta il Governo utilizza i progetti di legge e i decreti-legge come *spot* pubblicitari, annunci su ciò che farà, sugli obiettivi che vuole conseguire; ma poi queste norme non vengono attuate, o vengono modificate prima della loro attuazione, così come nel caso di alcune norme contenute in questo decreto-legge rispetto alle disposizioni già approvate con la legge finanziaria. Ancora una volta devo ribadire e rilevare con rammarico che la Carta delle autonomie locali non è stata approvata. Non se n'è neppure iniziato l'*iter* parlamentare. Manca pertanto un quadro organico di riordino delle competenze degli enti locali, del loro assetto istituzionale. Questa Carta doveva essere approvata già prima della legge sul federalismo fiscale, perché dava il quadro istituzionale su cui poi innestare le norme di carattere fiscale e finanziario. Non è stato fatto. Vi è stato l'impegno del Governo e del ministro Calderoli a dare immediatamente avvio al suo *iter* legislativo e invece ora, ad un anno ormai di distanza dall'approvazione della legge sul federalismo fiscale, il testo è appena stato depositato dal Governo alla Camera. Camera. Nel merito, si tratta di un decreto-legge contenente materie estremamente eterogenee, che assembla aspetti finanziari e ordinamentali, in evidente contrasto con i presupposti di necessità ed urgenza che l'articolo 77 della Costituzione prevede prevede come indispensabili per la decretazione d'urgenza. È un decreto-legge che si caratterizza per una logica di forte centralizzazione, che è peraltro uno degli elementi caratterizzanti la politica di questo Governo. Il Partito Democratico ha più volte sostenuto - e il disegno di legge che abbiamo presentato, a mia prima firma, sulla carta delle autonomie locali lo dimostra che è indispensabile percorrere tutte le strade e tutti i processi che evitino gli sprechi causati dalla ridondanza e dalle duplicazioni degli assetti istituzionali e organizzativi. Riteniamo che sprecare risorse nelle strutture e nelle sovrastrutture significhi ridurre le risorse per i servizi essenziali per i cittadini, per la qualità della loro vita e delle città e per la qualità dell'ambiente. Siamo veramente sicuri, colleghi senatori, che siano la riduzione di alcuni consiglieri provinciali e comunali, di qualche assessore e la soppressione degli ATO o del difensore civico comunale le scelte decisive per il risparmio e per la riduzione degli sprechi? Non pensiamo che queste norme attengano in modo diretto alla democrazia, alla possibilità stessa di avere una rappresentanza, anche per le forze politiche non particolarmente ampie? Non ci accorgiamo che, mentre facciamo queste scelte, alziamo la soglia di ingresso per la rappresentanza delle forze politiche in queste istituzioni locali? E poi si tratta di norme invasive dell'autonomia istituzionale, statutaria ed organizzativa degli enti locali, autonomie garantite dalla Costituzione.

che ha fatto dell'autonomia e del federalismo a parole, sbandierato ma non praticato, la sua bandiera appunto. Alcune considerazioni nel merito di una norma, che ritengo importante ma che non posso condividere, così come è stata definita, la norma relativa al Patto di stabilità. Ritengo che sia giusta la riduzione della rigidità e dei vincoli del Patto di stabilità, in particolare con riferimento alle risorse che provengono agli enti locali in modo diretto ed indiretto dall'Europa, fondi europei che sono indispensabili nelle politiche di formazione e di sostegno allo sviluppo economico ed alla coesione sociale; fondi che se non vengono spesi in un tempo determinato, debbono essere ristornati all'Unione europea. Credo che questa sia una scelta giusta, ma non credo che sia altrettanto giusto togliere dal vincolo del Patto di stabilità tutti - dico tutti - i grandi eventi. È vero che è giusto non penalizzare i Comuni e le Province coinvolti nei cosiddetti grandi eventi ma basta leggere l'elenco di quei 45 grandi eventi, per i quali sono state fatte le ordinanze della Protezione civile, per comprendere con chiarezza che non si tratta di iniziative così grandi, così rilevanti e soprattutto così prioritarie. Allora, il Partito Democratico indica, rispetto al Patto di stabilità e alla riduzione dei suoi vincoli, altre scelte davvero maggiormente prioritarie, in particolare quelle relative alla sicurezza delle scuole e all'edilizia scolastica, per cui il Governo ha promesso, ma non lo ha mai messo a disposizione concretamente, un miliardo di euro. Penso alla sicurezza ambientale, alle opere di rilievo sociale per gli anziani e i disabili, alle infrastrutture. Ci sono tanti, tanti investimenti che possono essere molto più prioritari, capaci di essere realizzati con grande rapidità e quindi anche in grado di sostenere l'occupazione e lo sviluppo economico.

Ed è la strada di definire l'assetto delle autonomie locali e le loro competenze, superando la frammentazione di queste competenze, le loro duplicazioni o triplicazioni perché in questo caso, sì, che si tratta di sovrapporre delle spese, anche inutili, solo di carattere strutturale. Individuiamo la strada di assottigliare le strutture dei Ministeri, sia a livello centrale sia a livello territoriale, in corrispondenza della devoluzione di funzioni. Rimane sempre tutto inalterato al centro e credo che invece sia necessario assottigliare le strutture centrali.

infine, se il Governo vuole proprio chiedere un ulteriore sforzo e un ulteriore impegno alle autonomie locali - voglio ricordare che proprio Comuni e Province hanno maggiormente contribuito, molto di più delle strutture centrali e nazionali, alla riduzione dell'indebitamento e della spesa pubblica -,

una quota da destinare all'assetto istituzionale ed ordinamentale ed alle spese inerenti al funzionamento delle strutture. Chiedo in una parola al Governo di dire se nelle autonomie crede o non crede; se delle autonomie si fida o non si fida; la smetta allora di incidere proprio su di loro per ottenere la maggior parte dei tagli sulla spesa pubblica.

Ovviamente non potevamo che adottare e portare avanti il criterio che avevate ormai stabilito, con questo gioco un po' perverso del trasferimento dallo Stato agli enti locali; avremmo voluto l'altro processo, che era molto più trasparente e chiaro,

fondamentale per la nostra comunità e la montagna in particolare; ridà spazio e centralità agli enti locali e alle Regioni per quanto riguarda il Patto di stabilità; un controllo delle spese e delle indennità dei nuovi consigli regionali; fa, quindi, economia a tutti i livelli. Ovviamente, siamo pronti in qualsiasi momento anche a intervenire a livello centrale. Presidente, vorrei brevemente richiamare l'ordine del giorno G106, che chiede al Governo di intervenire per confermare e specificare ulteriormente, ove fosse necessario, che tra i contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, devono ritenersi esclusi i contributi erogati dallo Stato a valere sul fondo sviluppo investimenti qualora questi siano utilizzati dagli enti locali nelle infrastrutture per quanto riguarda il servizio di tipo integrato. Ora non è così: gli ATO non riconoscono queste spese sostenute dagli enti locali, ledendo quindi anche la capacita di investimento degli enti locali.

che conferma questa interpretazione. Chiediamo che il Governo la ribadisca, liberando importanti risorse per gli enti locali e facendo giustizia, come vorrà sicuramente fare, per quanto riguarda il territorio.

del decreto-legge in titolo, ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime sul testo, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni: con riferimento all'articolo 4, commi 4 e 4-*septies*, il ricorso alle risorse del fondo ordinario di cui al capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, pone profili problematici sul piano del sistema contabile, posto che nel momento attuale dell'esercizio finanziario non appare determinabile l'ammontare delle risorse sovrabbondanti sul suddetto capitolo, atteso che la garanzia in ordine alla sussistenza di tali risorse è connessa all'effettivo accertamento delle stesse alla fine dell'esercizio a seguito delle necessarie certificazioni da parte degli enti locali; inoltre, si osserva che il ricorso alle risorse del fondo ordinario di cui al capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno in questione, poste che le stesse sarebbero destinate ad andare in economia a fine esercizio, costituisce una metodologia che appare critica sul piano della correttezza contabile; si osserva altresì che alla luce del ricorso alle risorse in questione si pongono profili critici in ordine alle modalità di costruzione dei tendenziali di spesa, risultando necessario operare una riflessione sul piano metodologico circa i criteri adottati per il rispetto dei criterio della legislazione vigente. Il parere è altresì reso, con riferimento all'articolo 3, nel presupposto che l'indennità massima prevista come riferimento per la retribuzione dei consiglieri regionali sia considerata in senso stretto, senza ricomprendere diarie, rimborsi spese o qualsiasi altra corresponsione corrisposta ai membri del Parlamento. In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti

Esprime poi parere di nulla osta sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.20, 1.48, 1.49, 1.55, 3,4,

che ove uno di tali emendamenti fosse approvato in relazione ad ogni singola tipologia di copertura il parere è da intendersi contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui restanti. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti».

cessa questa confusione, sospendo la seduta. Non sono in grado di annotare i pareri del Ministro!

Il Governo, con questo comma, si è disinteressato delle montagne, ed è anche andato oltre definendo, con un comma della finanziaria, che il criterio di montanità

tutti i Comuni montani (e non solo a quelli definiti precedentemente). Si tratta però di briciole. Non è un progetto, ma è una mera distribuzione, senza che per la montagna emerga un vero progetto di *governance*. Le comunità montane hanno svolto, e stanno svolgendo, un importante ruolo, uno sviluppo dei territori, sia delle Alpi che degli Appennini. Si è data, finora, dignità a questi territori, che faticano a tenere il passo con i ritmi

1-*quinquies*, introdotto dalla Camera dei deputati nel testo originario, che stabilisce, a mio giudizio in maniera eccessivamente semplice e *tranchant*, l'attribuzione alle Regioni per la rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali. Con questo ordine del giorno si vuole sollecitare il Governo a far sì che tale rideterminazione avvenga nel rispetto non solo degli obiettivi di tutela ambientale, ma soprattutto delle prerogative costituzionali dei Comuni, e che questa rivisitazione, sempre ai fini del contenimento della spesa pubblica, possa stabilire nuove dimensioni territoriali, anche a scavalco dei confini amministrativi perché, soprattutto per quanto riguarda gli ambiti idrici, il rispetto

deriva anche da una previsione della finanziaria del 1998 che ha istituito un particolare regime di tesoreria restrittivo per i grandi Comuni e per le Province con popolazione superiore ai 400.000 abitanti.

se vogliamo ridurre il debito pubblico nel suo complesso, credo ne abbiamo l'opportunità attraverso l'erogazione delle somme bloccate dal 1998 presso le tesorerie centrali. erogare queste somme a condizione che vengano impegnate quali avanzi di amministrazione per la riduzione del debito degli enti locali. Tutto questo farebbe un buon servigio agli enti locali e soprattutto un grande servigio al debito pubblico nella sua totalità.

delle prerogative del Parlamento da parte del Governo. Poiché si tratta di una materia molto delicata ed importante, e visto che il ministro Calderoli ha avuto la cortesia di interloquire su questo punto,

i seguenti emendamenti concernenti i rinnovi elettorali anticipati e i requisiti di eleggibilità per le elezioni amministrative: 1.46, 1.47, 1.0.1 e 2.0.1. deroghe particolari al Patto di stabilità: 4.57, 4.63, 4.78, 4.81, 4.82; 4.39, 4.40, 4.52, 4.54; 4.300, 4.301, 4.302, 4.303, 4.304; 4.53; 4.60 e concernenti agevolazioni in favore di determinati enti locali e categorie: 3.4; 4.47, 4.48, 4.49; 4.98, 4.100; emendamenti concernenti imposte, tributi e tasse di interesse locale: 4.87, 4.0.15; 4.24, 4.0.1, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.14; 4.0.17, 4.0.18, 4.0.19, 4.0.20, 4.0.21; 4.19 concernenti il patrimonio immobiliare degli enti locali: 4.89, 4.0.8, 4.0.9 e 4.0.10.

sono presenti in tribuna gli alunni della Scuola media «Ugo Foscolo» di Perugia. A loro va il saluto dell'Assemblea.

**Il Senato non approva.**

Dal momento che è diffusa la consapevolezza della opportunità di trattare in maniera differenziata i servizi idrici rispetto ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, noi potremmo accettare di trasformare gli emendamenti in ordine del giorno, confermando la volontà del Governo, nella modifica del decreto legislativo n. a trattare in maniera differenziata i servizi pubblici locali attinenti alle gestioni idriche e prevedendo che le concessioni di captazione, derivazione e accumulo della risorsa idrica per usi potabili vengano assegnate alla esclusiva titolarità di soggetti pubblici di governo, definiti dagli enti locali. Con questo contenuto noi possiamo ritirare gli emendamenti trasformandoli in ordine del giorno.

mi sembra utile porre l'accento sulla necessità della chiarezza di cui i nostri enti locali devono disporre nell'applicare la normativa. Già abbiamo una normativa sui servizi pubblici locali, in particolar modo per quanto riguarda l'acqua, confusa, non sempre chiara e di non immediata interpretazione; ora l'abolizione degli ATO - gli ambiti territoriali ottimali - sebbene condivisa, senza un riferimento immediato in ordine a chi vadano attribuite quelle competenze, può ingenerare ulteriore confusione nel territorio, ulteriori difficili interpretazioni e ulteriori ricorsi legali. L'emendamento 1.300 è il tentativo di ridurre questa confusione e di ricondurre le competenze oggi assegnate all'ATO nell'alveo dell'amministrazione provinciale, previa anche l'attivazione di una consultazione degli enti locali. per rispetto degli enti locali stessi, che nell'ambito di questa legge appaiono spesso mortificati. Penso che la gestione dei servizi pubblici, in particolar modo la gestione dell'acqua, debba essere prima di tutto dell'ente locale. l'emendamento va nella direzione di riportare le competenze degli ATO esattamente nell'ambito degli enti locali invece di affidarle genericamente ad una competenza regionale, sapendo che oggi gli enti locali rischiano di essere mortificati, oltre

Presidente, questo nostro emendamento mira a

di servizio: mi riferisco specialmente al Nord Italia ed ai Comuni amministrati dalla Lega. Non si capisce perché non possiamo abolire questa norma, che è appunto una forzatura che nulla ha a che vedere con quello che ci richiede l'Europa, fermarci un attimo per stabilire quali sono i criteri per poter assicurare un servizio che garantisca l'acqua come bene pubblico - diritto di tutti - e che quindi ne garantisca l'accesso a tutti, ma altresì la qualità, un uso sostenibile dal punto di vista ambientale e ne riduca gli sprechi che in questo Paese sono drammatici. Credo che così facendo, con estrema laicità, si uscirebbe

dal punto di vista della qualità del servizio offerto e delle tariffe che crescono, e via dicendo. Quindi, se accoglieste questo nostro emendamento, abolendo quella norma

quei gestori che non garantiscono il servizio di qualità necessario, quindi facendo un servizio al Paese. Per questo vi invito a votare a favore di questo emendamento,

Signor Presidente, signor Ministro, voglio ricordare ai colleghi che circa un anno fa la Commissione affari costituzionali ha iniziato l'esame dei disegni di legge presentati da alcuni Gruppi parlamentari in materia di codice delle autonomie. Il Presidente della Commissione affari costituzionali, senatore Vizzini, coerentemente con quello che fu l'orientamento anche nella scorsa legislatura, ha assegnato il compito di relatori a due colleghi, uno della maggioranza e uno dell'opposizione; è quindi iniziato un esame molto attento di un di un provvedimento che riveste particolare importanza. L'esame della Carta delle autonomie si è poi fermato perché la Commissione ha deciso, su impulso della maggioranza e su una pressione molto forte del Governo, di affrontare prima il tema del federalismo fiscale. Abbiamo sostenuto in quella sede con grande convinzione - e ne siamo convinti oggi più che mai - che si è trattato di un primo e grave errore. Che senso ha, colleghi, discutere del modo con cui devono essere distribuite le risorse senza avere prima discusso seriamente chi fa che cosa, cioè quali sono le attribuzioni e le funzioni degli enti locali? Ma poiché la maggioranza del centrodestra, in particolare la Lega, avevano assoluta necessità di alzare la bandiera del federalismo fiscale, così è stato. In quest'Aula, in occasione dell'approvazione del disegno di legge sul federalismo fiscale, a cui i Gruppi di opposizione e, segnatamente, il Partito Democratico, hanno dato un contributo di grande rilievo,

autonomie. Dall'approvazione di quel disegno di legge sono passati alcuni mesi e tale provvedimento, nel frattempo approvato dal Governo dopo una lunga gestazione, è stato assegnato alla Camera dei deputati che ne ha iniziato daccapo l'esame. Devo dire, Devo dire, francamente, che su questa sottrazione e su questo scippo al Senato della Repubblica abbiamo protestato in modo energico, non per difendere le prerogative del Senato ma per l'esigenza di investire la Camera che più aveva lavorato su questo argomento. Il disegno di legge giace quindi in questo momento in Commissione senza che sostanzialmente ne sia iniziato l'esame. Nel frattempo, Presidente, e questa è la cosa più grave, il Governo interviene nella materia del codice delle autonomie per esempio sul numero e la composizione dei consiglieri comunali, sulle municipalità di quartiere, sui consigli regionali: questioni certamente delicate, che sono l'oggetto

Così è avvenuto anche in questo campo; durante l'esame della legge finanziaria, è stato inserito un intervento legislativo che ha inciso profondamente, suscitando grande preoccupazione e vibrate proteste nel mondo delle autonomie per quanto riguarda la composizione dei consigli comunali, di municipalità e di quartiere. Oggi il Governo è stato costretto a fare una vigorosa marcia indietro.

costituzionali del nuovo Titolo V e lo facciamo con interventi al contrario, che vengono inseriti ora in un decreto-legge ora in una finanziaria; ci si rende poi conto due mesi dopo che si è sbagliato clamorosamente e si ricomincia da capo.

sottoporre alla vostra attenzione che questo modo di legiferare è profondamente errato,

sull'eliminazione delle cause di ineleggibilità per coloro che fanno parte di enti diversi e a sancire una volta per tutte che le dimissioni, al fine di poter essere candidati e quindi eletti,

il senatore Mercatali, volto ad affrontare il tema del Patto di stabilità interno. Approfitto di questo intervento, signor Presidente, perché rimanga agli atti che, a mio giudizio, alcune dichiarazioni di improponibilità

che riguarda il Patto di stabilità interno esattamente negli stessi termini con cui se ne parla all'interno della norma in questione. Pertanto, nel giro di 15 giorni, siamo passati da dichiarazioni di improponibilità che che - in un contesto nel quale c'era l'esigenza di essere assai laschi - sono state secondo me troppo generose nei confronti dei proponenti, ad una situazione nella quale, siccome bisogna approvare il testo così com'è, le dichiarazioni di improponibilità hanno uno spettro a mio giudizio decisamente troppo ampio. In ogni caso, per quanto riguarda specificamente l'emendamento 4.29, il Patto di stabilità interno,

ha due fondamentali difetti. Il primo è che esso è "stupido", per usare un aggettivo che l'ex Presidente del Consiglio dei ministri impiegò con riferimento al Patto di stabilità europeo. Perché il Patto di stabilità interno, così com'è, è stupido? Perché non presenta il carattere di flessibilità necessario per consentire agli enti locali, soprattutto sul lato della spesa in conto capitale,

Questo è un difetto gravissimo in una situazione come quella che noi stiamo vivendo, nella quale avremmo bisogno, come dell'aria da respirare, esattamente dalla possibilità di consentire tenere rigorosamente sotto controllo la spesa corrente, ma di avere una politica di bilancio espansiva per realizzare quegli investimenti di cui l'economia e la società italiana hanno drammaticamente bisogno per rendere la crisi meno pesante e anche meno duratura. Il secondo difetto del Patto di stabilità interno è il suo carattere chiaramente lesivo dell'autonomia degli enti locali. Il

nella gestione del Patto di stabilità interno nel loro rapporto con i rispettivi enti locali. Ora, a questo a questo proposito, nella legge di contabilità così come da noi definita nella lettura al Senato (e poi modificata alla Camera), avevamo introdotto una regola a mio giudizio particolarmente interessante. Essa voleva, contemporaneamente, rendere il Patto di stabilità interno meno stupido (nel senso di cui ho già detto) e soprattutto meno rigido, affidando alle Regioni un'attività di programmazione e di gestione tale per cui i Comuni potessero scambiarsi tra di loro titoli di debito, a seconda della situazione economica e delle decisioni di investimento che i diversi Comuni volevano prendere.

di gestire molto più flessibilmente, sulla base della programmazione regionale, la loro finanza. Quel testo è stato eliminato ma noi tendiamo, almeno in parte, a riproporre attraverso questo emendamento

la fornitura di beni o servizi, adesso non le possono pagare perché, altrimenti, violano il Patto di stabilità interno. Mi rivolgo ora ai colleghi che vantano la loro esperienza di amministratori locali. Chiunque faccia l'amministratore locale sa che sono oggi decine i Comuni che si trovano in questa situazione. Si tratta, quindi, di una manifestazione particolarmente grave della stupidità del Patto, alla quale ho già fatto riferimento.

crisi è determinata non dalla scelta delle banche, ma dalla scelta della pubblica amministrazione (in particolare del sistema delle autonomie locali) di non pagare in tempo. Le amministrazioni locali, però, non possono pagare in tempo perché, altrimenti, violano il Patto

sulla pubblica amministrazione un obiettivo flessibile di risparmio e si utilizza questo risparmio per finanziare la flessibilizzazione del Patto di stabilità interno. Si interviene poi con tagli lineari alla spesa,

si decidesse a fare propria quest'impostazione, forse si potrebbe contemporaneamente lavorare alla riforma della pubblica amministrazione e ad interventi contro la crisi che abbiano un minimo di efficacia. *(Applausi dal

Signor Presidente, intendo illustrare l'emendamento 4.66, che propone la soppressione del comma 4-*novies*.

favorevoli a prevedere norme di maggiore flessibilità, che consentano in modo particolare agli enti locali di far fronte alle esigenze di investimenti infrastrutturali, per la messa in sicurezza delle scuole e del territorio, coprendo le maggiori esigenze finanziarie che in questo modo si verrebbero a determinare attraverso interventi altrettanto penetranti, che attualmente non si fanno, sui Ministeri centrali, considerato che in questi anni la spesa a livello centrale è paurosamente aumentata ed è totalmente fuori controllo. Si è invece operato in modo particolarmente penalizzante sugli enti locali, anche al di là di qualunque ragionamento circa il peso effettivo della spesa locale sulla spesa complessiva della pubblica amministrazione allargata.

in esame si introducono due abnormità ulteriori. La prima riguarda il fatto che si induce ad eccessivamente, fuori da ogni logica, le ordinanze di protezione civile e si insiste lungo una strada sbagliata, già oggetto di dura sanzione e discussione anche in questa sede e su cui si è riusciti ad ottenere qualche modifica; ma questa norma dimostra che il Governo è recidivo, nel senso che vuole ulteriormente andare lungo la via di una deroga costante alle norme di buon funzionamento della pubblica amministrazione. La seconda abnormità sta nel fatto che si inducono i Comuni a dichiarare grande evento o, per meglio dire, a chiedere la dichiarazione di grande evento per poter sforare i limiti del Patto di stabilità interno. Proprio per evitare queste assurdità e abnormità, chiediamo all'Aula di votare a favore di questo emendamento soppressivo.

*(PD)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 4.77 che vuole modificare la disposizione inserita nella finanziaria per il corrente anno, la quale prevede di trarre risorse dai beni della Difesa per ripianare i debiti del Comune di Roma. Il decreto in esame conferma quella disposizione e cerca di evitare il giudizio di incostituzionalità che la minaccia, considerate le precedenti decisioni della Suprema corte, istituendo una Conferenza dei servizi nell'ambito della quale gli enti locali approverebbero la destinazione d'uso dei beni militari. Rimangono dubbi sul fatto che questa norma possa superare le obiezioni. Ma l'aspetto più grave sta nel fatto che la costituzione di fondi di investimento per reperire risorse da destinare al Comune di Roma rappresenta un precedente rischioso dal punto di vista politico e amministrativo. Ancora una volta un testo del Governo si rivela un buon affare per gli investitori che parteciperanno ai progetti, ma non per la struttura statale interessata che in questo caso, tra l'altro, ha urgente bisogno di risorse finanziarie, a causa dei consistenti tagli che sono stati apportati negli ultimi due anni al suo bilancio. In sostanza, in un momento in cui le nostre Forze armate sono fortemente impegnate in Italia e all'estero, è incredibile che esse debbano rinunciare ai loro immobili, talvolta anche preziosi, senza ottenere benefici finanziari che possano almeno in parte compensare quei drastici tagli. Benefici finanziari che sono in realtà indispensabili per migliorare le condizioni di vita del personale e il funzionamento delle strutture; per mantenere in servizio i volontari in ferma prefissata, hanno operato con professionalità in Italia e all'estero e che dovranno invece lasciare l'uniforme; per confermare quelle capacità operative dei reparti, che hanno consentito alle Forze armate italiane di farsi apprezzare in tutti i teatri operativi del mondo. Riteniamo quindi necessario intervenire con l'emendamento di cui prima parlavo, chiedendo che almeno una quota non inferiore al 25 per cento del valore degli immobili ceduti sia destinata alla Difesa. Se l'emendamento non sarà accolto, la Difesa subirà purtroppo una penalizzazione che non merita, e ciò avverrà sicuramente per scarsa considerazione da parte di chi è preposto all'economia del Paese, ma anche per insufficiente attenzione e tutela da parte di coloro che frequentemente esaltano l'importanza delle nostre Forze armate, in realtà però solo a parole e non concretamente nei fatti. Signor Presidente, il parere è ovviamente contrario a tutti gli emendamenti presentati. Vorrei soffermarmi però sulla questione del Patto di stabilità, sollevata dai senatori Il Patto di stabilità è sicuramente criticabile per molti aspetti; in ogni caso, dovrà essere rivisto con il passaggio al federalismo, perché dovrà essere adottata una regola molto più semplice quella del pareggio del bilancio, tagliando in tal modo la testa al toro. Tutto sommato, però, nella sua stupidità, tale Patto persegue l'obiettivo di far sì che il nostro Paese adempia agli obblighi del Patto di stabilità europeo

Allora, è chiaro che spendere di più potrebbe avere una funzione anticiclica (chi lo nega?): però, spendere di più oggi significa avere più debiti domani. E abbiamo presente la situazione di altri Paesi europei che si trovano in quella condizione. La domanda è: ce lo possiamo permettere? se guardiamo la ripartizione complessiva della spesa pubblica e il funzionamento del Patto, non è vero che gli enti locali abbiano avuto una penalizzazione maggiore rispetto al contenimento della spesa previsto per altri livelli di governo o per altri tipi di enti pubblici. Questo perché, in fondo, è vero che gli enti locali sono enti autonomi, ma l'autonomia non è qualcosa che in qualche modo premia rispetto al diritto generale dei contribuenti ad essere colpiti il meno possibile. Quindi, l'autonomia è

Gli enti autonomi è giusto che siano autonomi, ma l'autonomia è un valore non in assoluto, ma sempre relativo rispetto ad un obiettivo di carattere più generale. Il

sugli altri emendamenti dichiarati improponibili, pur essendo opinabile, in alcuni casi, il giudizio della Presidenza. Non l'abbiamo fatto perché in altre occasioni

semplicemente ignora precise richieste provenienti dalle opposizioni. A nome del Gruppo le ho avanzato la richiesta precisa di pronunciarsi, prima di procedere al voto sugli emendamenti riferiti all'articolo 4,

Man mano che andiamo avanti con gli emendamenti, quando lei riterrà che un emendamento faccia riferimento a questo pacchetto ne discuteremo. Mi sembra una procedura ragionevole.

Mauro Maria Marino, Sanna, Vitali, Carloni, Giaretta, Legnini, Lumia, Lusi, Milana, Morando, Nicola Rossi, Barbolini e Marcenaro, chiedo a 15 colleghi di appoggiare la richiesta per poter procedere alla votazione elettronica.

Vitali, Carloni, Giaretta, Legnini, Lumia, Lusi, Milana, Morando, Nicola Rossi, Barbolini e Marcenaro, chiedo il sostegno a 15 colleghi per poter esprimere il voto mediante

fatto riferimento con molti emendamenti per contribuire a risolvere un problema affrontato dal Governo in modo un po' raffazzonato da molto tempo a questa parte. Su tale emendamento, che porta la firma dei senatori Bianco, Mercatali, Adamo, Bastico. Ceccanti, De Sena, Incostante, Mauro Maria Marino, Sanna, Vitali, Carloni, Giaretta, Legnini, Lumia, Lusi, Milana, Morando, Nicola Rossi, Barbolini, Marcenaro, con l'aggiunta della senatrice Pignedoli, che mi ha chiesto di rivolgere

*(PD)*. Signor Presidente sull'emendamento 4.15 a firma dei colleghi Sanna, Mercatali, Bianco, Adamo, Bastico, Ceccanti, De Sena, Incostante, Mauro Maria Marino, Vitali, Carloni, Giaretta, Legnini, Lumia, Lusi, Milana, Morando, Nicola Rossi, Barbolini, Marcenaro e a cui hanno chiesto di aggiungere la firma la senatrice Armato e i senatori Garaffa e Pegorer,

Il vice ministro Vegas ha sostenuto, a ragione, la necessità assoluta di avere un patto di stabilità interno. Se noi non legassimo con il patto di stabilità interno la finanza dello Stato centrale a quella del sistema delle autonomie autonomie non saremmo in grado di rimanere all'interno dell'area dell'euro perché non saremo mai in grado di rispettare il Patto di stabilità e di crescita che ci lega ai nostri partner. Il punto è che il Patto di stabilità interno, che è certamente necessario, può essere meno stupido di quanto non lo sia oggi. E al riguardo credo, peraltro, che il vice ministro Vegas Abbiamo avanzato proposte, che il Vice Ministro conosce, non per eliminare il Patto di stabilità interno, che riteniamo tanto necessario quanto lo ritiene necessario il Governo, ma per correggerlo in alcuni dei suoi aspetti qualificanti. In secondo luogo, il vice ministro Vegas ha sostenuto che spendere di più da parte del sistema delle autonomie locali avrebbe oggi una funzione anticiclica positiva a causa della situazione di crisi nella quale siamo precipitati, ma significherebbe anche, inesorabilmente, secondo il vice ministro Vegas, aumentare il deficit ed il debito e, quindi, esporre il Paese a rischi sotto questo profilo. Su questo punto non siamo d'accordo, non perché pensiamo che occorra aumentare il deficit e il debito, ma per la ragione esattamente opposta. La nostra proposta cioè consentire, agli enti locali di poter spendere di più se sono enti locali virtuosi che rispettano il Patto di stabilità interno e sono in grado oggi di sostenere una spesa in conto capitale, che svolgerebbe una positiva una positiva funzione anticiclica. Tale proposta verrebbe coperta inoltre con riduzione di spesa corrente primaria, che, come è noto, ha un livello di capacità di svolgere una funzione anticiclica decisamente inferiore rispetto alla spesa in conto capitale. In ultimo, approfitto della dichiarazione di voto per dare un suggerimento al Governo. Il Vice Ministro potrebbe trovare ben 80 milioni di euro - non una cifra

80 milioni di euro sono destinati, mediante quel comma 13 dell'articolo 2, ad un fantomatico ente locale di cui alla legge finanziaria del 2006

Ebbene, siamo andati a verificare qual è l'ente locale. Si tratta del Comune di Roma: c'era da aspettarselo, ma adesso lo sappiamo. Tutta quella tiritera relativamente alla «legge di cui...» serve solo a non scrivere nella norma Comune di Roma. Roma. Abbiamo cercato poi di capire quali sono gli adempimenti comunitari che il Comune di Roma deve fare e per i quali riceve la bella sommetta, *ope legis*, di 80 milioni di euro.

fiscali, considerate aiuti di Stato illegittimi, alle società che gestiscono servizi pubblici locali a prevalente capitale pubblico. In conseguenza di quella decisione della Commissione europea, le società a prevalente capitale pubblico che gestiscono servizi pubblici locali hanno dovuto pagare nel 2009 - lo sapete, perché ce ne siamo occupati in occasione dell'esame di un decreto lo scorso anno

importanti società a prevalente capitale pubblico, che gestiscono bene servizi pubblici locali, hanno dovuto pagare 600 milioni di

dei Comuni non hanno distribuito dividendi nel 2009 o, se li hanno distribuiti, lo hanno fatto in quantità molto minori rispetto al passato. È risultato, un grave danno per il bilancio dei Comuni di Milano, Roma, Genova, Torino, Padova, Verona, Venezia, Brescia, e potrei continuare

del vostro principio di rispetto dell'autonomia locale! Se il Governo vuole trovare 80 milioni di euro da concedere al sistema delle autonomie per fare fronte meglio, ad esempio, ad una politica di investimenti pubblici prenda quegli 80 milioni e li distribuisca a tutti i Comuni d'Italia, anche a quello di Roma, ma *pro quota*.

Presidente, preciso la richiesta di riammissione di alcuni emendamenti perché i numeri non sono consecutivi e quindi non vorrei che ne omettessimo qualcuno.

riammesso una serie di emendamenti perché, nel momento in cui si approva un provvedimento che riguarda interventi urgenti concernenti gli enti locali, non si capisce perché non si affronti in maniera adeguata la questione del Patto di stabilità. Mi soffermo su un punto che riguarda una questione molto delicata, in particolare i lavori pubblici degli enti locali. Si diceva prima che se

Se solo si sbloccassero, si compirebbe un intervento di carattere straordinario che sicuramente darebbe una risposta significativa a una serie di imprese e di aziende che operano L'altra questione riguarda la messa in sicurezza del territorio. Noi continuiamo a prestare attenzione all'emergenza e agli interventi di emergenza e non mettiamo un euro per la prevenzione

Presidente, stiamo proponendo diverse soluzioni positive, costruttive, anticicliche ed utili al Paese sul Patto di stabilità interno. Con tale emendamento su cui penso il Governo dovrebbe meditare e cambiare idea rispetto al parere negativo che ha formulato e su cui la stessa maggioranza potrebbe convenire. C'è un modo moderno C'è un modo moderno di agire nella lotta alla mafia: responsabilizzare i Comuni, farli diventare un elemento dirompente e positivo in grado di colpire gli interessi mafiosi ed il sistema delle collusioni, che spesso si annidano a livello locale, tanto da infiltrare le amministrazioni e fare dei danni incalcolabili alla legalità,

per la promozione dell'associazionismo antiracket e per il risanamento dei quartieri ad alto disagio sociale. Una moderna frontiera è quella di saper coniugare a livello locale legalità e sviluppo; a livello locale, nei Comuni,

e quindi bisogna ristrutturarli. Spesso ciò non è possibile; in qualche caso diventa anche un alibi, ma in moltissimi casi per molti Comuni, anche virtuosi, è impossibile utilizzare e destinare gli investimenti per tale nobilissima e modernissima finalità.

e, quindi, avere un sostegno della comunità locale a questa scelta dirompente. Immaginatevi ancora se in molti Comuni dove - adesso anche al Nord, ad esempio Milano - c'è una penetrazione territoriale delle mafie

premia i Comuni virtuosi e mette finalmente in un dinamico rapporto contro le mafie la dimensione della legalità con quella dello sviluppo locale. Penso che una proposta di questo tipo vada accolta e la ribadiremo quando parleremo nei prossimi giorni di agenzia sui beni confiscati, perché lì vi chiederemo che una parte del cosiddetto fondo per la giustizia

impattano con un patto di stabilità stupido e incoerente e, quindi, non viene data loro la possibilità di utilizzare eventualmente una norma che premi i Comuni che vogliano investire in una moderna scelta antimafia.

Desidero solo consegnare alla Aula qualche riflessione in merito, auspicando da parte del rappresentante del Governo un qualche chiarimento, in quanto la vicenda - com'è noto - com'è noto - discende da una sentenza pronunciata nel luglio scorso dalla Corte costituzionale, la n. 238, la quale ha riconosciuto la natura tributaria della tariffa dell'igiene ambientale, ponendo due grandi problemi. luogo la necessità di un intervento normativo che porti chiarezza in materia, perché la Corte ha certificato l'esistenza di un problema, ma tocca al Governo e al Parlamento dare risposte risolutive alla questione.

però, nonostante l'imbarazzo e l'ammissione che il problema esiste, abbiamo ascoltato solo generici impegni e parole consolatorie. Il problema è che adesso le scadenze vengono a rogito e il 30 aprile è una data che incombe. Il 30 aprile ci saranno delle conseguenze. Abbiamo provato a suggerire con l'emendamento 4.0.16 un percorso che sostanzialmente interpretasse la necessità di normare, senza creare però sconquassi.

fattore IVA all'interno della tariffa ci saranno imprese - ad esempio nei distretti industriali - che si vedranno applicare una quota di esercizio della prestazione maggiorata che non potranno scaricare perché non è più una tariffa, ma un tributo. Secondariamente, ci saranno Comuni che, dovendosi riprendere in carico la gestione diretta di questa attività, avranno disagi di

che si tratta di 1.300 Comuni su 8.000 - non sono bruscolini - che hanno il merito di avere, prima di altri e con difficoltà, applicato norme di legge e che sono stati, per questo, beffati due volte: quando hanno dovuto ristrutturare i loro bilanci perché venivano meno alcune entrate pagando in termini di Patto di stabilità e quant'altro, ed oggi, perché dovranno sostenere ulteriori costi e conflittualità con i cittadini nel rapporto e nella relazione con l'erogazione di questi servizi. Trovo questa situazione incomprensibile e non capisco perché i tanti amministratori presenti all'interno della maggioranza e tra le file della Lega si ostinino a non considerare e a non prendere sul serio un problema che genererà difficoltà di funzionamento nei Comuni, disagio nei cittadini, incomprensione nelle imprese, con ciò soprattutto contraddicendo le tanto conclamate dichiarazioni secondo le quali si vuole premiare il merito, la correttezza amministrativa e la serietà di chi fa bene l'esercizio della sua responsabilità.

Infatti, se i problemi possono essere affrontati in una sede più familiare e più vicina alla gente come è l'amministrazione comunale,

Vengo pertanto alle principali osservazioni sull'impostazione generale di questo disegno di legge che, licenziato dalla Camera con l'ennesimo ricorso al voto di fiducia sul maxiemendamento presentato in Aula dal Governo, arriva in Senato per essere approvato in pochissimi giorni a causa della sua imminente scadenza, addirittura pochi giorni prima delle elezioni regionali. In questo modo, la maggioranza ha di nuovo svuotato il Parlamento delle sue prerogative, facendolo apparire agli occhi degli italiani un'istituzione inutile, con l'obiettivo di esaltare il mito del Governo del fare: a Palazzo Chigi si lavora, alla Camera e al Senato, al contrario, si perde tempo o al massimo si ratifica. Al contrario, il provvedimento avrebbe meritato un maggiore dibattito e un più ampio confronto, se solo la maggioranza avesse dimostrato un minimo di coraggio riformatore. Esso invece rappresenta l'ennesima occasione persa di questo Esecutivo per dare una risposta compiuta ed organica ad alcuni dei problemi percepiti come urgenti dai cittadini, in quanto loro particolarmente vicini: la riforma degli enti locali. Con questo disegno di legge si concretizza invece una disciplina frammentata, frutto di una procedura priva di confronto preliminare con le autonomie locali. Stiamo discutendo di modifiche che intervengono sulla legge finanziaria approvata da questo Parlamento appena due mesi fa: dunque, siamo in presenza di una legislazione occasionale, casuale - per così dire - e scoordinata. Al contrario, sarebbe stato opportuno definire una disciplina organica e corrente della materia. Avremmo potuto esaminare in primo luogo il codice delle autonomie, al fine di affrontare la questione in una cornice complessiva e in un'ottica di sistema. Anche alla luce dei recenti avvenimenti giudiziari, vi è una forte e comprensibile esigenza del Paese di una maggiore etica nella pratica delle amministrazioni statali, a tutti i livelli di governo. Si chiede di ridurre i costi della politica, di rendere più efficienti ed efficaci i controlli e meno clientelare la pubblica amministrazione. A tale proposito, siamo completamente d'accordo con l'obiettivo che persegue il disegno di legge, anche se non è sempre conforme ai principi che mi sono permesso di elencare. A questa serie di drammatiche richieste si risponde pertanto solo parzialmente, con la riduzione dei costi della politica, ma anche con la riduzione della democrazia stessa. Infatti, a fronte di risparmi irrisori, dovuti al taglio di un certo numero di consiglieri comunali, si registra l'ulteriore riduzione degli spazi per i consiglieri nominati. Ciò significa che vi saranno ancora meno controlli, perché i consigli comunali, attraverso la dialettica tra maggioranza e minoranza, rappresentano la prima forma di controllo sugli atti delle giunte, mentre gli assessori o i dirigenti non eletti non rispondono ai direttori, ma solo a chi ha dato loro l'incarico. Faccio una piccola parentesi su quelle autonomie locali

eliminerà praticamente l'unico consigliere italiano presente. Pertanto, anche da questo punto di vista vorremmo esprimere la nostra preoccupazione. Oggi nel Paese vi è una forte e giustificata esigenza di dare una spinta alla nostra economia incagliata nella crisi. Le imprese hanno bisogno di liquidità per non essere costrette a licenziare, le famiglie hanno bisogno di reddito per non ridurre ancora i consumi. Questo provvedimento di cui discutiamo non è lo strumento adeguato per rendere meno rigida l'interpretazione del Patto di stabilità interno per i Comuni, anzi peggiora la situazione, se si tagliano ulteriormente i trasferimenti di risorse agli enti locali, non si sa come si potranno gestire le amministrazioni comunali nei prossimi anni. Eppure in Italia abbiamo Comuni che hanno in cassa le risorse per spendere, per rilanciare quelle piccole e grandi opere infrastrutturali che dovrebbero dare lavoro a migliaia di piccole e medie imprese. Sono soldi che servirebbero a rimettere in moto l'economia e l'occupazione e invece vengono tenuti bloccati, congelati in attesa di non si sa che cosa. Questa è una dimostrazione che sul federalismo le idee sono ancora molto confuse e non tutti lo percepiscono come era stato espresso nel disegno di legge da noi tutti approvato, che si baserebbe sul principio della sussidiarietà. Intanto, vengono

quelli che non hanno debito ed anzi hanno risorse disponibili che però vengono paralizzate, allora ancora una volta si dà la sensazione di usare due pesi e due misure. Dobbiamo dare risposte concrete anche ai servizi pubblici locali. È necessario dare risposte per consentire la sopravvivenza di molti Comuni che sono il cuore e il motore dell'economia nazionale e delle politiche sociali. Abbiamo bisogno, pertanto, non di un disegno di legge parziale, ma di una riforma organica che risponda all'esigenza di autonomia degli enti locali, che dia forza all'associazionismo attraverso le unioni di Comuni e che, soprattutto, risponda seriamente alle esigenze dei cittadini e della nostra comunità. Non vi è dubbio che bisogna razionalizzare e ridurre i costi degli organi dell'indirizzo politico e degli enti locali regionali e limitare, conseguentemente, le spese degli apparati a quelle strettamente necessarie accrescendo, al contempo, la trasparenza, la responsabilità dell'agire amministrativo con la finalità ultima di rafforzare il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni. facciamolo in maniera efficace, tenendo in mente la necessità che la riforma generalmente invocata assuma finalmente carattere organico.

annuncio il voto di astensione del nostro Gruppo.

si va affermando e consolidando una prassi per la quale i decreti-legge vengono esaminati con grande fretta e, si direbbe, quasi a scatola chiusa in Commissione. Anzi di più: il presente provvedimento, data la sua imminente scadenza, non è stato esaminato affatto nel merito in Commissione e, solo sommariamente, in Assemblea. Di fatto, l'apodittica enunciazione da parte del Governo dell'esistenza delle ragioni di necessità e di urgenza riferite ad un provvedimento normativo travolge in un solo colpo il principio costituzionale del bicameralismo paritario (il decreto è stato velocemente esaminato soltanto dalla Camera dei deputati), oltre che i Regolamenti parlamentari (il decreto è stato esaminato soltanto dall'Assemblea). Chiederei un po' di silenzio, signor Presidente, perché il Gruppo Italia dei Valori intende, con la sua dichiarazione, precisare una posizione importante sul piano politico. Nel merito del provvedimento, sotto il profilo generale, ci si trova dinnanzi ad una sorta di schizofrenia normativa deducibile dalla presentazione di una serie di provvedimenti, da parte del Governo, vertenti sulla medesima materia, ma che recano contestualmente disposizioni tra loro in gran parte disomogenee e divergenti. È deplorevole poi il metodo utilizzato dal Governo che, per l'ennesima volta, si concretizza in una disciplina frammentata e disomogenea, in una procedura priva di previo confronto con le autonomie locali. Sarebbe stato quanto mai opportuno definire una disciplina della materia organica e coerente trasferendo il contenuto del decreto-legge in esame nell'ambito del disegno di legge di riforma delle autonomie locali, già all'esame della Camera. Il provvedimento, nella sua parte finanziaria, tocca maggiormente le difficoltà che i Comuni e gli enti locali in generale stanno attraversando; gli enti locali sono gli unici che hanno contribuito e stanno contribuendo al tentato risanamento dell'assetto della finanza pubblica: nel 2008 hanno ridotto il loro indebitamento netto di oltre 1,2 miliardi di euro, con ulteriori 300 milioni nel 2009. Un elemento di fortissima criticità per gli enti locali è rappresentato dalle disposizioni relative al Patto di stabilità interno. Il famoso decreto-legge n. 112 del 2008 ha, infatti, fissato un contributo per il comparto Comuni, per il risanamento della finanza pubblica, molto elevato, creando rilevanti difficoltà nella gestione della cassa per gli investimenti. Il Governo ha poi dovuto correggere il tiro, sia pure parzialmente, con due decreti-legge nel corso del 2009, che hanno dato la possibilità ai Comuni di escludere dal Patto alcuni pochi pagamenti per gli investimenti. Si doveva, viceversa, escludere dal computo dei saldi validi ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno le spese per gli investimenti dei Comuni virtuosi, finanziando così opere pubbliche di piccole e medie dimensioni, immediatamente cantierabili, adatte all'intervento delle piccole e medie imprese. Si sarebbe creato certamente un volano per le attività economiche, con un effetto di traino tanto più prezioso in questa fase di crisi economica e occupazionale, tenendo anche conto che le spese degli enti locali per le opere pubbliche rappresentano più del 60 per cento delle spese in conto capitale delle nostre pubbliche amministrazioni. Oppure, considerato il precario equilibrio creatosi dopo la crisi finanziaria che ha colpito il nostro Paese, sarebbe stato utile fornire ai Comuni uno strumento, già presente nella legge n. 311 del 2004, che consentisse di anticipare le spese in conto capitale finanziate antecedentemente al 2009 a carico di un fondo appositamente istituito presso la Cassa depositi e prestiti. In ogni caso, sarebbe stato necessario non penalizzare i Comuni che autonomamente hanno adottato nel 2009 misure atte a sostenere l'economia in un momento di forte crisi come quello attuale, contribuendo al sostegno dei lavori pubblici di piccola e media entità; ciò ha prodotto effetti anticiclici sull'economia locale e nazionale positivi e sui livelli di occupazione delle imprese più deboli. Importanti misure sono state adottate da parte di molti Comuni anche sul versante della spesa destinata al sociale; ciò al fine di minimizzare le ripercussioni della crisi economica sulle fasce più deboli della popolazione. Per questo sarebbe stato opportuno - come peraltro richiesto dall'ANCI - sospendere per il 2009 l'applicazione delle sanzioni previste dai commi 20 e 21

Con un emendamento dei relatori alla Camera - perché qui, ricordo, non abbiamo esaminato un bel niente! - si è prevista l'esclusione dal saldo finanziario di tutte le entrate e le spese sostenute dai Comuni in attuazione di ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri destinate a fronteggiare emergenze o grandi eventi come l'Expo di Milano. Stesso ragionamento sarebbe stato opportuno fare per le risorse provenienti dai vari Ministeri destinate a prevenire disastri naturali controllabili, quali ad esempio il dissesto idrogeologico, fronteggiato con apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Ma il Governo non ha sentito ragioni, impegnato com'è a definire leggi e leggine per risolvere i guai giudiziari del *Premier*, invece di occuparsi seriamente di risolvere i problemi dei cittadini comuni. Sono da due anni ormai che è così. Anche sul fronte della riduzione dei costi della politica locale sono stati fatti grandissimi *spot* con mediocri risultati. Cerco di dimostrarlo. Lo *spot*: la finanziaria 2010 stabiliva che i Comuni dovessero dal 2010, man mano che si rinnovavano i consigli, ridurre del 20 per cento il numero dei consiglieri, mentre il numero massimo degli assessori doveva essere ridotto ad un quarto dei consiglieri stessi; le Province dovevano avere un numero massimo di assessori pari ad un quinto dei consiglieri. Parliamo, quindi, di oltre 160.000 poltrone locali che subivano una sforbiciata di notevole entità. Inoltre, i soli Comuni dovevano, obbligatoriamente, provvedere ad una serie di misure con la soppressione dei difensori civici e la soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale. Questo era lo *spot*. La realtà: con il decreto-legge al nostro esame, rimane immutata la riduzione dei trasferimenti ordinari nel triennio 2010-2012, ma si allontana di un anno - e poi vedremo - lo sfoltimento degli organi della rappresentanza locale. Secondo la modifica introdotta dal decreto-legge in esame, per l'anno 2010 la riduzione dei trasferimenti è spalmata su tutti gli enti locali (Comuni e Province). Tale decisione conferma l'assoluta mancanza di concretezza del Governo Berlusconi che agli annunci non fa seguire fatti inoltre, finisce con il colpire i servizi dei Comuni (il taglio riguarda trasferimenti di parte corrente) e così il nocumento si estende, evidentemente, ai cittadini contribuenti. Questi fatti, cari colleghi, ci fanno dubitare fortemente delle reali intenzioni del Governo di procedere con convinzione sulla strada della riduzione dei costi impropri della politica. In definitiva, la questione finanziaria degli enti locali sta davvero diventando drammatica. Lo stanno toccando con mano gli amministratori, siano essi di centrosinistra o di centrodestra, e lo stanno soprattutto toccando sulla loro pelle i cittadini, perché i tagli che sono stati fatti agli enti locali, e in particolare ai Comuni, sono quelli che vanno ad incidere più direttamente e pesantemente sui cittadini: mi riferisco, in particolare, agli odiosi tagli sulle politiche sociali e assistenziali, alle politiche della casa, alle risorse per gli asili nido. I tagli fatti all'inizio della legislatura e l'eliminazione dell'ICI hanno messo gli enti locali letteralmente in ginocchio. È vero che con questo decreto si sono razionalizzate le composizioni dell'apparato politico degli enti locali, ma probabilmente bisognava procedere con più coraggio

«Se uno il coraggio non ce l'ha, non se lo può dare». Per questi motivi, che riguardano questioni sia di metodo parlamentare che di merito legislativo, dichiaro, a nome del Gruppo parlamentare Italia dei Valori, il voto convintamente contrario al disegno di legge in oggetto. *(Applausi

è opinione condivisa da parte di tutto il nostro Gruppo che il percorso fatto per questo decreto-legge sia stato esauriente e approfondito, in modo particolare nell'altro ramo del Parlamento. È un altro passo verso quell'azione riformatrice a cui la Lega Nord tiene molto. E noi siamo anche molto convinti che affrontare i problemi che riguardano il nostro Paese con impegno e serietà, caro senatore Barbolini e colleghi dell'opposizione, ed è quello che noi cerchiamo di fare. Ma, come avete visto, non abbiamo raccolto nessuna delle vostre provocazioni fatte oggi e indirizzate, in modo particolare, al Gruppo Lega Nord. Dico solamente e semplicemente che si potrà fare meglio, si potrà fare di più, ma oggi abbiamo iniziato a fare questo che è importante. A questo proposito vogliamo anche dare atto all'opposizione del contributo offerto nel coniugare l'azione di contenimento della spesa all'utilità delle amministrazioni locali. Forse è solo un dettaglio, che però appartiene

voteremo contro questo provvedimento per una ragione principale: è un provvedimento che va nella direzione contraria a quella che servirebbe per una seria riforma federalista. Signor Ministro, noi possiamo accettare che i tempi della riforma federale siano molto più lunghi di quelli che avevate promesso in campagna elettorale o al momento dell'approvazione della legge sul federalismo fiscale. Non ci sfuggono i complessi nodi politici e tecnici che condizionano la realizzazione di un assetto federale: politici, perché alla fine si tratta di togliere risorse ad una parte degli enti locali per premiare gli enti locali più virtuosi; tecnici perché, ad esempio, individuare in modo corretto il caposaldo dell'assetto della procedura federalistica, che è il costo *standard*, non è semplice. Signor Ministro, da noi non sentirà mai su questi punti una critica populistica o retorica, quel tipo di critica che non manca mai sulle labbra del Presidente del Consiglio. Semmai, troverà un sostegno quando si trattasse di procedere seriamente sulla strada della realizzazione del federalismo fiscale. Quello che non possiamo accettare è che le nuove leggi siano centralistiche e rinneghino alle radici gli orientamenti necessari lungo la strada del federalismo. Che federalismo è quello che ci proponete con questo provvedimento? Chiedete ai Comuni di risparmiare e i risparmi vanno allo Stato che non sa risparmiare. Bisognerà pur dire, infatti, che in questi ultimi due anni la spesa per i consumi intermedi dello Stato, che ritrae abbastanza esattamente quello che serve per far funzionare lo Stato centrale, è aumentata nel 2008 di 6,4 punti e nel 2009 di altri 7,5 punti. Lo Stato amministrato da voi costa molto di più: la spesa dello Stato centrale cresce molto di più dell'inflazione e molto di più del PIL Insomma, è un federalismo che toglie ai Comuni per dare allo Stato. Nel 2011, a regime, questo insieme di risparmi dovrebbe dare un gettito di 86 milioni di euro, e di tanto avete tagliato e taglierete i trasferimenti ai Comuni.

Il Comune di Roma viene ristorato di un evento fiscale che ha portato a una minore distribuzione di dividendi da parte delle società ex municipalizzate, ma come questo Comune ce ne sono decine che hanno subìto lo stesso danno. Un solo Comune viene premiato

riceveranno dei beni demaniali in stato di degrado, spenderanno un mucchio di soldi per poterli manutenere e non incasseranno nemmeno l'ICI che prima lo Stato pagava ai Comuni per quei beni. È questo il federalismo che volete? Noi pensiamo che si potrebbe fare molto di più, in attesa del federalismo che verrà: premiare l'accorpamento dei Comuni, incentivare sul serio le gestioni associate, vincolare in modo particolare i Comuni maggiori a una solida *spending* *review* dei propri bilanci, rafforzare i meccanismi premiali e punitivi per la buona e la cattiva spesa. Di tutto questo purtroppo non c'è nulla. Vi è però un secondo aspetto che desidero mettere in luce. Quale disegno istituzionale sul ruolo delle assemblee democratiche locali emerge da questo provvedimento? Badiamo bene, le assemblee democratiche locali sono state il presidio della democrazia nel nostro Paese: la vitalità della democrazia in Italia cammina sulle gambe della ricchezza della rappresentatività a livello delle singole comunità locali. Nei consigli comunali si è formata la classe dirigente politica del Paese e forse dovremmo riflettere sul fatto che uno dei motivi dell'inefficienza crescente del sistema di funzionamento delle istituzioni centrali è che si è reciso questo rapporto tra la politica locale e la politica centrale. Pensate davvero che sia decisiva qualche centinaia di consiglieri comunali in meno nel nostro Paese, la maggior parte dei quali svolgono un lavoro puramente volontario di rappresentanza degli interessi della cittadinanza? Perché, mentre tagliate i consiglieri comunali (ripeto, in gran parte persone che fanno volontaristicamente il loro lavoro), intanto aumentare a dismisura gli apparati dello Stato centrale. Portateci qui le tabelle dei dipendenti e dei consulenti della Presidenza del Consiglio e di pezzi di Stato privatizzati,

si faccia un passo in avanti per il nostro Paese? Noi pensiamo di no. Tra queste cose che qui ci proponete e una solida ambizione di un riformismo federale non c'è veramente nessuna parentela, e per questo motivo voteremo dunque convintamente contro. *(Applausi dal

Onorevole Presidente, colleghi, deluderò chi è ansioso di ascoltare un lungo e diffuso intervento; lo so che me lo richiedete, ma vi deluderò.

introduzione vorrei semplicemente rilevare che il Governo ha preso l'iniziativa e si è assunto la responsabilità, con decreto, di far entrare in vigore alcune norme che anticipano il disegno del codice delle autonomie e alcune altre che concretizzano invece interventi immediati ispirati alla contingenza, apparsa meritevole di essere affrontata con questo primo pacchetto di misure non rinviabili. Ebbene, il nostro Gruppo condivide con il Governo l'analisi che sta alla base del provvedimento, la prima selezione di temi e snodi sui quali si è deciso di intervenire, l'entità degli interventi e delle previste ricadute funzionali e finanziarie. questa, in sintesi, è appunto la ragione politica per la quale, complessivamente valutata, la conversione in legge riceve ora il nostro voto favorevole. Nel corpo della dichiarazione, a cui rimando, traccio un quadro dello scenario delle ipotesi di riforma complessiva sia dei governi locali sia delle istituzioni parlamentari e di Governo, nonché di quelle regionali, che rappresentano anche nella nostra visione aspetti di unico palinsesto meritevole di una profonda azione riformatrice, passo in esame i passaggi essenziali di questo provvedimento, che, con luci ed ombre, sotto taluni aspetti, ma con ombre necessitate da quella che era appunto la ragione fondante dell'intervento, riscuotono complessivamente la nostra convinta adesione. Si conclude questa mia dichiarazione con un auspicio di carattere politico. L'auspicio conclusivo (ho scritto e dico) tanto più conferente, se proviene da noi che sosteniamo il Governo e questo suo provvedimento, è che tutta la materia delle autonomie dedotta in progetti di riforma trovi un sistematico approfondimento in questa Camera, a prescindere da quale ramo del Parlamento ne sia prioritariamente investito, poiché i Gruppi intendono sicuramente assumere ponderatissime responsabilità nel varare riforme destinate